*(Segue la verifica del numero legale)*. Il Senato è in numero legale.

L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

notizia di pochi minuti fa la scomparsa, all'età di novant'anni, di Dario Fo, che è stato un grande protagonista della cultura italiana, europea e mondiale del nostro tempo, insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1997. Dario Fo, attore, autore e regista, ha innovato profondamente il teatro comico italiano e la nostra letteratura attraverso spettacoli realizzati spesso insieme alla moglie Franca Rame, che fu anche componente di quest'Assemblea nella XV legislatura. Paradigmatico dei motivi ispiratori e della sua produzione teatrale in generale è l'opera «Mistero buffo» del 1969, una rielaborazione di antichi testi popolari della tradizione lombarda con continui innesti della cultura contemporanea e continui riferimenti alla vita civile e sociale del nostro tempo. Dario Fo fu un intellettuale fortemente impegnato in campagne politiche e civili significativa è, a questo riguardo, la motivazione dell'assegnazione del premio Nobel: «Perché,» - diceva quella motivazione - «seguendo la tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi». Il Senato della Repubblica si unisce quindi al dolore della famiglia e di tutti gli italiani per la scomparsa di un grande artista e intellettuale. Invito pertanto l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

*(PD)*. Signora Presidente, vorrei chiedere cortesemente ai colleghi

non mi è mai interessato sapere cosa votasse Dario Fo, quale scheda inserisse nell'urna; so soltanto che con Dario, un uomo scomodo,

Per chi lo ha conosciuto, come me, e ha avuto l'onore anche della amicizia sua e della carissima Franca, che abbiamo ricordato anche in questa

la stagione delle bombe a Milano, piazza Fontana, il suo impegno incessante, i suoi spettacoli teatrali alla Palazzina Liberty. Per più di una generazione è stato un punto di riferimento nel modo di vedere la realtà, nella capacità di non essere conformisti. Venne cacciato dalla RAI, dal servizio pubblico, perché si era permesso, in una sigla di «Canzonissima», di parlare contro la guerra e di mettere in evidenza le vedove delle guerra, queste donne lasciate sole dall'orrore della morte. Venne cacciato, ma andò avanti e fece teatro. Fu amato indipendentemente dai mezzi di informazione,

Aveva una cultura artistica straordinaria e una capacità di divulgazione davvero molto rara. Era un grande studioso di linguistica e il «Mistero buffo» ne faceva una sorta di Rabelais contemporaneo. Ricordo lo studio sulla lingua e la sua capacità di rendere un dialetto progressivo, ma assolutamente comprensibile a tutti; perché, come sempre, nel teatro, oltre alla parola, c'è il gesto e, oltre al gesto, c'è la presenza scenica, c'è quella empatia che lui sapeva trasmettere a tutti. Ci mancherà tantissimo questo valore artistico molto particolare. Quando vinse il premio Nobel non ci credeva neanche lui, aveva timidezza e ritrosia: e ritrosia: era contento e preoccupato al tempo stesso di avere una responsabilità così grande. Ne abbiamo parlato alcune volte e lo capisco, come capisco la sua lontananza progressiva dal mondo dopo la scomparsa della sua amatissima Franca, che è stato un pezzo della sua vita e di se stesso. Credo che dopo la sua morte sia iniziato un declino - ahimè che è comune a tutti gli uomini, ma che quando si verifica anche per la mancanza di amore, per la perdita della persona che si ama, sia ancora più forte. Ci sarebbero da dire moltissime cose e spero che potremo farlo in quest'Aula con una celebrazione adeguata ad un premio Nobel, oltre alle nostre povere e piccole parole; indispensabili, però, perché quando muore

Non si rassegnava al passare del tempo. Era un eterno ragazzo e la trasgressione era la sua vita. Persino quando venne candidato sindaco da una lista civica in un Consiglio comunale, fece un programma stranissimo, complicatissimo e impossibile da realizzare. Era però la sua cifra; quell'impossibilità che poteva trovare soluzione e spazio soltanto nell'arte, in quell'arte straordinaria che lui ci ha lasciato e che ci fa sentire un pochino più soli tutti quanti oggi, e che spero potremo insieme condividere per tanto e tanto tempo, insegnandola ai più giovani. L'arte del teatro è infatti la vita e credo che noi tutti, in un periodo così orribile e complicato, abbiamo bisogno di sentire l'arte e la cultura come l'unico vero antidoto ai fondamentalismi, agli egoismi,

Presidente, anche noi siamo costernati dalla notizia del decesso di Dario Fo, questo genio di

unici nel panorama del mondo attuale, di cui egli ha compreso le contraddizioni e

l'apprezzamento da parte della cultura liberale quale noi esprimiamo, è un apprezzamento di grande coerenza nel senso che l'uomo libero nel mondo deve essere messo nelle condizioni di esprimere all'infinito tutte le sue potenzialità. Per quanto riguarda la storia della persona, è stato qui accennato alla RAI. Per alcuni versi, è stato anche l'anticipatore di una contestazione, del modo paludato di fare intrattenimento e spettacolo nella RAI. Tanto è vero, come è stato qui ricordato, ne fu cacciato. È stato anche l'anticipatore e l'antesignano di quella posizione presa poi dal principale *competitor* della RAI, che è stato Silvio Berlusconi nel fondare il sistema Mediaset. Mediaset. Al pari di Berlusconi, infatti, lui ha messo in discussione quel sistema paludato e quel sistema anche curiale di trattare lo spettacolo ed anche l'informazione. Addirittura Berlusconi ne è stato anche oggetto di sberleffo, come del resto era nel DNA del personaggio. Da questo punto di vista anche il suo

Grazie, presidente

Tuttavia, egli va sicuramente ricordato come grande uomo di teatro. Egli stesso, ricevendo il premio Nobel, che gli fu dato con le motivazioni che la signora Presidente ha ricordato, disse: «Con me hanno voluto premiare la gente di teatro». Fu infatti un caso anomalo che un autore più che altro di testi teatrali e, in primo luogo, un attore di testi teatrali ricevesse il premio Nobel. Come tale si è comportato, in modo simile a tanti altri uomini d'arte, in particolare del teatro, teatro, rappresentando un pungolo, un feroce contrappunto al potere - come scrissero coloro che gli hanno assegnato il premio Nobel - ma soprattutto alla parte politica politica di volta in volta a lui avversa. Questo fatto lo ha messo sulla stessa posizione di altri grandi uomini di teatro. uno tra i tanti, Aristofane, che era pungolo anche per alcuni che poi sono diventati dei mostri sacri: il grande nemico di Aristofane era infatti Pertanto, anche in quel caso c'era una parte politica avversa ad un'altra. In questo Dario Fo ha avuto un'irruenza, un'esuberanza e un coraggio, che lo hanno portato ad assumere posizioni estremamente discutibili. Credo che non si possano tacere - come non si dovrebbero tacere a proposito di altri intellettuali della nostra storia recente - le sue posizioni riguardanti il commissario Calabresi,

con grandi capacità teatrali, con grande irruenza e con la capacità di farsi ascoltare da un pubblico molto vasto, pur praticando un genere teatrale che poteva

gran parte della fama di Dario Fo, questo personaggio avverso al potere - come lo definì la commissione che assegnò il premio Nobel - così scomodo, con posizioni estreme, assolutamente avverso all'area

ne uscì di sua volontà - e in parte a ciò spinto - per poi rientrarvi non molti anni dopo, negli anni Settanta. Credo che questa vicenda ci debba ricordare che anche la RAI di oggi dovrebbe poter dare spazio a qualcuno che naturalmente abbia delle capacità,

Io spero che questo possa succedere anche oggi, benché di fatto spesso non accada. La testimonianza di Dario Fo la ritengo positiva in questo senso: aver saputo mettere alla prova quel potere, potere, un potere democratico che ha dato spazio anche a lui che gli era radicalmente e violentemente avverso. Temo che bisognerebbe

Presidente, credo che fossimo tutti impreparati alla morte di Dario Fo, perché certi vecchi che sono sopravvissuti alla storia del nostro Paese, a loro stessi, a tanti amici, alle *élite* che li hanno confortati hanno confortati e accompagnati, a un certo punto ci sembrano immortali, ci sembra che non possano mai morire. A nome nel Gruppo vorrei fare le condoglianze a Jacopo Fo, che continua il lavoro del padre.

premio Nobel: «Seguendo la tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi».

il compiacimento di un artista che vedeva riconosciuto un ruolo non comune della cultura. Dario non era

Abbiamo parlato di politica con Dario Fo; lui ascoltava, non sparava sentenze, ma in ogni momento rivendicava il diritto dell'artista di essere in qualche modo anarchico,

una battaglia di interpretazioni, spaccando il capello, dicendo cosa fosse giusto e cosa non lo fosse, cosa si poteva fare e quale critica fosse eccessiva, perché questa critica fondata nello studio della grande tradizione nazionale era fondamentale per il potere. la senatrice Franca Rame, con la sua lettera di dimissioni parlò, forse prima del tempo, di una cosa che tutti voi senatori avete constatato - vi piaccia o meno - in questa legislatura: della crisi d'identità fortissima

Era una RAI ossessivamente democristiana, perché venivamo da una crociata: le elezioni del 1948, con la scomunica dei comunisti e dei sindacalisti, erano state una crociata; era però una RAI che apriva a tutti, che aveva moltissimi intellettuali comunisti nel suo gruppo di comando. Ed era capace di coinvolgere quella straordinaria *élite* milanese che non era solo Dario Fo. Penso a Walter Chiari, ma anche a Enzo Jannacci. C'erano un sacco di uomini di teatro e di spettacolo particolarmente vitali

accennato sulle pagine dei giornali tra Scalfari e Zagrebelsky: certo che esistono le *élite,* i numeri uno non esistono se non sono in qualche modo connessi con le *élite*. Quella RAI onnivora sapeva mettere tutto dentro, ma naturalmente bisognava stare nel limite

e che stentava ad aprire al centrosinistra negli anni Sessanta. Ora, credo che a Dario quella espulsione dalla RAI abbia fatto uno straordinario favore e piacere. Dario si è messo a studiare. «Mistero buffo» è una delle opere magnifiche magnifiche degli ultimi cinquant'anni: la cultura popolare italiana che diventa teatro, critica corrosiva, arte pura. La sua partecipazione ai tumultuosi eventi successivi, quelli del Sessantotto, è un atto di testimonianza e di critica. Così come un atto di testimonianza e di critica è stata la sua simpatia, nell'ultimo periodo, per il Movimento 5 Stelle, nel quale vedeva una voglia di rinnovamento molto forte, al di là dei capelli che si spaccano, delle posizioni che possono essere sbagliate o della critica che può essere populista. Come ebbe a spiegarmi, e gliene sono ancora grato, quando mi disse: «Guarda, c'è una realtà della politica e poi c'è una realtà della storia. E nella realtà della storia noi

altro da dire, così a braccio, ma spero che lo commemoreremo come merita, senza dire troppe cose formali e lasciandogli la sua

Signora Presidente, per noi è semplicemente morto un corpo, perché il suo spirito aleggia in ognuno di noi, che gli abbiamo voluto un gran bene e lo ricordiamo semplicemente con il suo sorriso e il suo affetto. In ogni momento ci ha sempre detto: non mollate. Egli è semplicemente una persona libera. Non sarebbe mai entrato in un luogo come quest'Aula. E anche sua moglie, Franca Rame, non vedeva l'ora di andare via da questo luogo

così, semplicemente, con un saluto, un ringraziamento e un abbraccio di affetto. Un affetto infinito che non si conclude adesso, né si potrà mai concludere. E lo ringraziamo per tutto ciò che ci ha insegnato, sia come persone, sia come cittadini, sia come popolo. Grazie. Grazie, Dario.

Presidente, tenuto conto dell'ordine del giorno e di come i lavori si stanno sviluppando, chiedo all'Assemblea l'inversione dell'ordine del giorno, anticipando la discussione dei disegni di legge

Ogni sette secondi si sposa una bambina con meno di quindici anni. Già questi dati, presentati da Unicef e Save the children in occasione della Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze martedì scorso, basterebbero per capire l'importanza della mozione che votiamo oggi. Ma lo scenario in realtà è ancora più grave. Bambine e ragazze, costrette a sposarsi, abbandonano la scuola rinunciando quindi al principale strumento di *empowerment* personale, di autonomia e anche di arricchimento della società, visti i numerosi studi che collegano l'aumento del tasso di scolarità al PIL. Bambine e ragazze obbligate ad accettare matrimoni precoci devono poi subire le proposte sessuali dei mariti, con gravidanze precoci e rischi per la salute, sia delle bambine madri che dei bambini. Così 70.000 ragazze ogni anno muoiono per le complicazioni durante gravidanza o parto e i bimbi che nascono da una madre minorenne hanno il 60 per cento in più di probabilità di morire ancora neonati. Se sopravvivono, poi, rischiano più degli altri di soffrire di denutrizione e di ritardi cognitivi o fisici. I matrimoni precoci sono diffusi in diversi contesti politici e culturali, soprattutto nell'Asia meridionale e nell'Africa subsahariana; non a caso le stesse aree in cui sono maggiormente diffusi mortalità materna e infantile, malnutrizione, analfabetismo. Lo voglio dire con chiarezza: non si tratta, però, di un fenomeno connesso solo alla povertà,

prima delle battaglie e delle vittorie delle donne, anche nella nostra società le bambine erano poco incoraggiate a studiare, destinate a lavori in casa e spesso costrette a matrimoni di convenienza. Da noi le cose sono per fortuna cambiate e stanno cambiando, ma non ancora in altri contesti. Dobbiamo allora attivarci maggiormente, informando, sensibilizzando, mobilitando le coscienze, mostrando la nostra vicinanza e adottando misure legislative e piani specifici di cooperazione nei Paesi dove queste pratiche ancora esistono e, contemporaneamente, operare in Italia. Anche perché, in particolar modo con l'incremento dei flussi migratori dai Paesi arabi e dal subcontinente indiano la presenza delle comunità straniere nelle nostre città, il matrimonio precoce coinvolge anche chi vive nel nostro territorio. La responsabilità dell'accoglienza e dell'integrazione positiva ci sfida quindi anche su questo terreno: far conoscere a chi arriva da noi i diritti di cui può godere e fornire un sostegno reale da parte della nostra società e delle nostre istituzioni tutte sono fatti determinanti. Si tratta di una responsabilità nei confronti di chi arriva e di chi vive già qui da noi. Le bambine e le ragazze che crescono con noi, che frequentano le nostre scuole e che seguono percorsi di integrazione, finiscono spesso per allontanarsi, giustamente, dalle culture di provenienza, rifiutano i matrimoni combinati e si sentono così ancora più forzate violentate quando obbligate a sposarsi, rischiando di essere allontanate dalla comunità e di trovarsi senza assistenza, senza conforto e senza rapporti umani in cui rifugiarsi. È per loro, per ogni bambina e bambino che soffre e subisce violenza, in Italia e nel mondo, che dobbiamo, per le nostre responsabilità, agire. Vedete, il rispetto dei diritti umani di cui tanto spesso discutiamo deve sempre e ovunque essere una scelta e una

a svolgere il nostro ruolo da protagonisti su questa materia. Ecco perché la mozione di oggi. Ecco perché un intervento del Parlamento italiano, proprio pochi giorni prima della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, che si svolgerà il 20 novembre. Approvando la mozione, condivisa e sottoscritta da quasi tutti (ma penso che l'Assemblea produrrà un risultato importante per tutti), dobbiamo impegnare il Governo ad agire su tre fronti. Innanzitutto, è necessario attivarsi nelle sedi internazionali per garantire, in e più celermente, il pieno rispetto, da parte dei Paesi che ne sono firmatari, della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che anche noi abbiamo ratificato. Essa dispone che «gli Stati parte adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale - «per tutelare le fanciulle e i fanciulli contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, Sottolineo: «compresa la violenza sessuale», e un matrimonio forzato è violenza sessuale. È importante comprendere i concetti e i loro collegamenti. assumere, poi, tutte le opportune iniziative per la piena attuazione della risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che mette al bando i matrimoni precoci e forzati e quindi sollecita tutti gli Stati membri a emanare, applicare e rispettare, leggi e politiche volte alla prevenzione del matrimonio precoce e forzato e alla protezione dei soggetti a rischio, per garantire invece che il matrimonio si celebri unicamente con il consenso informato, libero e pieno dei coniugi. valutare, in uno scambio importante e sinergico con il Parlamento, l'opportunità di dotare l'Italia di un'apposita normativa per considerare reato il matrimonio forzato e tutte le attività ad esso connesse. pensiamo che il modello più avanzato sia quello della Svezia, che nel 2014 ha approvato una legge specifica, secondo la quale i minori non possono più ricevere autorizzazione a sposarsi prima dei diciotto anni e la pressione esercitata da genitori o parenti può portare ad una pena detentiva

I matrimoni precoci e forzati sono una grave violazione dei diritti umani, oltre che di ogni principio di civiltà, di libertà e di autodeterminazione della persona. Violano il diritto di bambine e ragazze di vivere con gioia, serenità e in piena e in piena autonomia. Impediscono di essere protagoniste della propria vita, di seguire inclinazioni e desideri, di innamorarsi e di scegliere liberamente quando creare una famiglia e di guardare con ottimismo al futuro. Tutte le bambine e tutti i bambini, invece, hanno diritto a crescere sereni e liberi di scegliere. Dobbiamo impegnarci su questo, su questo, a prevenire, oltre che contrastare, queste situazioni, i pregiudizi, le discriminazioni, le violenze e le diseguaglianze. In fondo, questi sono i nostri principi fondamentali di convivenza civile. Dobbiamo sentire davvero, e non solo a parole e non solo nelle giornate di celebrazione, il destino di ogni bambina e di ogni bambino d'Italia, in Europa e nel mondo, di ogni bambino che c'è e che nasce, dobbiamo restituire a tutte le bambine la possibilità di essere padrone del loro destino. Ne va del loro futuro, ma anche della dignità, della responsabilità e della convivenza civile di ognuna e di ognuno di noi. Per questo ringrazio tutte le firmatarie e i firmatari della mozione.

secondo il recente *dossier* "Indifesa" di "Terre des hommes" sulla condizione globale delle bambine e delle ragazze, ogni anno, circa 15 milioni di ragazze si sposano prima di aver compiuto i 18 anni. Tali dati sono destinati ad aumentare fino "ad arrivare a 950 milioni entro il 2030 e nel 2050 a un miliardo e 200 milioni di baby spose"; i Paesi in cui i matrimoni precoci sono maggiormente diffusi risultano essere: Somalia, Niger, Repubblica centrafricana, Mali, Sud Sudan, Guinea e Malawi. Si tratta di territori particolarmente fragili segnati da povertà estrema, guerre ed emergenze umanitarie. Sul punto, il Bangladesh è uno dei Paesi ove è più elevata l'incidenza dei matrimoni precoci: il 52 per cento delle adolescenti si unisce in matrimonio il 2 per cento ha meno di 11 anni; è di tutta evidenza che le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati colpiscono maggiormente i civili, in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici, violenze sessuali, sfruttamento, tratte, coercizione alla prostituzione, in un persistente quadro di aggravamento della violenza di genere, durante e dopo i conflitti; ulteriori fattori che elevano l'incidenza dei matrimoni precoci risultano essere le calamità naturali, quali: terremoti, alluvioni, cicloni; l'organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani, ha confermato numerosi episodi di rapimento da parte dei miliziani islamisti ai danni di bambini e bambine. Le bambine, nello specifico, non solo venivano costrette a lavori domestici forzati, ma venivano anche obbligate a subire abusi sessuali e a sposare i miliziani, in palese contrasto con i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la IV Convenzione di Ginevra, relativa Grazie, i dati dell'Islamic justice department di Amman (Giordania) rilevano come i matrimoni precoci rappresentino il 35 per cento del totale registrato tra i profughi siriani nel 2015. Il fenomeno, tuttavia, ha una maggiore estensione, in virtù del fatto che molte unioni non vengono registrate; la compravendita e la tratta di esseri umani, con particolare attenzione alle ragazze e alle giovani donne, rappresenta una delle più redditizie fonti per le casse del gruppo terrorista Stato Islamico. Secondo quanto riferito dall'Unami (United Nations Iraq), l'ISIS avrebbe aperto un ufficio a Mosul, istituendo un vero e proprio mercato, dove "le donne e le ragazze vengono esposte con cartellini dei prezzi, in modo che gli acquirenti possano scegliere e negoziare la vendita". Circostanze del tutto analoghe sono state segnalate anche Ramadi, a Falluja, così come ad Aleppo, Raqqa e al-Hasakhan. Città simbolo, queste, di un mercato in crescita, che si avvale in maniera strumentale delle nuove tecnologie. Le giovani ragazze e bambine, infatti, verrebbero vendute anche attraverso canali di messaggistica quali "WhatsApp" e "Telegram".

"Vergine. Bella, 12 anni. Il suo prezzo ha raggiunto i 12.500 dollari"; i flussi migratori hanno consentito l'affioramento di ulteriori evidenze. All'uopo, nel corso del 2015 il Dipartimento norvegese per l'immigrazione ha identificato 10 ragazze con

Nel febbraio 2016, il Ministro dell'immigrazione danese, a seguito dell'emersione di taluni casi, ha reso nota la volontà di bloccare l'accoglienza delle *baby* spose negli appositi centri. Diventare moglie in età precoce comporta pesanti ripercussioni sotto il profilo della salute nonché per l'armonico sviluppo psicofisico e sociale. Le bambine che vivono tale anticipata realtà, infatti, abbandonano prematuramente la scuola e sono costrette a gravidanze che il fisico non è in grado di affrontare e che le espone a gravi ed irreparabili conseguenze. Inoltre, la differenza d'età - spesso marcata - con il *partner* rende impossibile per le piccole spose di poter concordare l'uso di metodi contraccettivi, esponendole al rischio sia di contrarre malattie sessualmente trasmissibili, sia di gravidanze indesiderate, spesso molto rischiose. Sotto il profilo della natalità, ogni anno circa 16 milioni di ragazze aventi un'età compresa tra i quindici e i diciannove anni diventano madri, mentre è pari a circa un milione il numero di bambine con meno di quindici anni aventi la stessa sorte. Sono invece 3 milioni le ragazze aventi meno di vent'anni che hanno abortito in Paesi dove tale pratica è illegale o insicura. Sul punto, le complicazioni durante la gravidanza e il parto rappresentano, dopo i suicidi, la seconda causa di morte, con circa 70.000 ragazze che perdono la vita ogni anno. Inoltre, i bambini che nascono da madri adolescenti hanno il 50 per cento di probabilità in più di morire nei primi giorni dopo il parto, rispetto ai figli di donne tra i venti e i Si consideri che, ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la cosiddetta Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio». Inoltre, «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio». Si consideri anche che esiste una sempre più corposa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuclea rilevanti precetti per contrastare la violenza nei confronti delle donne.

consideri inoltre che, in data 22 ottobre 2014, in Commissione affari esteri alla Camera veniva approvata la risoluzione 7-00338, presentata dal Movimento 5 Stelle, a prima firma Maria Edera Spadoni, sul rispetto dei diritti dell'infanzia e delle donne in Iraq in riferimento alla questione delle spose bambine. In tale sede, il Governo si impegnava a «mantenere alta l'attenzione sul progetto di legge adottato dal precedente Governo iracheno ed ereditato dall'attuale Parlamento, anche in vista di possibili futuri passi che si si dovessero rendere necessari per impedire la sua eventuale adozione, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti e ratificati a difesa della dignità umana e dei diritti dell'infanzia e delle donne». Inoltre, in data 29 giugno 2016, presso il Consiglio d'Europa veniva presentata una mozione sul matrimonio forzato volta ad individuare misure necessarie alla sua prevenzione nonché all'identificazione di idonee metodologie, definizioni e criteri applicabili alla raccolta dei dati delle vittime di matrimoni forzati, in un'ottica di protezione delle vittime. In data 27 maggio 2014, la Svezia ha adottato un'apposita normativa volta a contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati,

Anzitutto, chiediamo che il Governo si impegni ad attivarsi, mediante l'utilizzo di ogni utile mezzo, presso le competenti sedi nazionali e internazionali, affinché siano compiuti tangibili passi volti al contrasto del fenomeno delle spose bambine, della violenza di genere contro le donne e dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i generi, soprattutto in via preventiva, mediante l'adozione di politiche efficaci e di concrete misure da attuarsi nei territori maggiormente a rischio, dando seguito ai precetti contenuti nella Convenzione di Istanbul e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; 2) ad assumere ogni necessaria azione, affinché si proceda, in tempi brevi, ad una compiuta raccolta, da parte degli organismi istituzionali, degli enti e delle organizzazioni competenti, dei dati inerenti al fenomeno delle spose bambine, nonché al successivo monitoraggio, studio, controllo, per ostacolare fattivamente tale ripetuta violazione dei diritti umani; ad incentivare, anche attraverso il coinvolgimento attivo delle organizzazioni internazionali governative e non governative riconosciute, un efficace piano di educazione ai diritti per le fasce di età maggiormente esposte,

delle donne, anche in tema di salute sessuale e riproduttiva, per il raggiungimento della parità di genere; 4) ad adoperarsi affinché, a partire dal contesto nazionale, ove si riscontra un vuoto precettistico, ogni Paese, attualmente inoperoso, implementi in maniera puntuale e cogente il proprio quadro normativo, mediante la previsione di specifiche fattispecie delittuose, sufficientemente sanzionatorie, sul matrimonio forzato; matrimonio forzato; 5) a garantire e a promuovere, anche negli idonei ambiti extraterritoriali, un'apposita protezione e la garanzia dell'anonimato a tutte le ragazze e le bambine che intendano denunciare reati e minacce,

a sostenere, anche nel contesto del dialogo e del confronto tra le nazioni in tema sanitario e di tutela dei diritti, nel caso di pericolo di vita della madre minorenne esposta a violenze e coercizioni e del feto, alla presenza di condizioni igieniche adeguate, il riconoscimento della pratica dell'interruzione di gravidanza,

il nostro Gruppo ha presentato una mozione in cui anche noi evidenziamo l'esistenza del drammatico fenomeno del matrimonio precoce, che vede bambine dall'infanzia negata, costrette a sposare uomini adulti e a portare avanti gravidanze in un'età in cui dovrebbero essere ancora figlie. Premesso che il matrimonio dovrebbe essere un momento importante nella vita di un individuo, un passaggio di crescita personale fondamentale e un impegno da assumere con responsabilità come base per la creazione di un famiglia, nel mondo è ancora drammaticamente diffuso il fenomeno del matrimonio precoce: bambine costrette a sposare uomini adulti e a diventare madri un'età in cui dovrebbero essere ancora figlie, con gravissime implicazioni sociali, psicologiche e sanitarie. I matrimoni precoci costituiscono, dunque, una violazione dei diritti umani.

poiché queste spose bambine sono vittime di violenze e soprusi e incapaci di prendere decisioni valide per loro stesse. Sul fronte dello sfruttamento, degli abusi e delle mutilazioni, i numeri sono altrettanto allarmanti. Dei 6,5 milioni di bambini tra i cinque e quattordici anni

Nei prossimi dieci anni, 30 milioni di bambine rischiano ancora di subire questa odiosa pratica. A fronte di un quadro del genere non è più possibile rimanere inerti. Bisogna porre fine a un tale vortice di violazioni di diritti, povertà, disuguaglianza, esclusione, coercizione, matrimoni forzati e gravidanze precoci, pressioni sociali e stereotipi Le bambine sono una porzione debole della nostra società; non possono difendersi, non hanno la forza e gli strumenti per ribellarsi al volere delle loro famiglie. Tocca quindi a noi aiutarle, difenderle, proteggerle, custodire la loro innocenza, garantire la possibilità di sognare un futuro con un uomo che scelgano liberamente. liberamente. Diverse Convenzioni internazionali, tra cui quella sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dalle Nazioni Unite nel 1989, obbligano gli Stati firmatari ad adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa al fine di tutelare i fanciulli da ogni forma di violenza,

affinché queste Convenzioni e risoluzioni internazionali vengano efficacemente rispettate. Poiché il fenomeno dei matrimoni forzati si sta registrando anche in Italia, a causa della presenza di molti immigrati, nella mozione chiediamo che si controllino gli stranieri che vivono in Italia per valutare se i matrimoni contratti coinvolgano o abbiano coinvolto minorenni e se, dunque, si possono ritenere frutto di violenza. di intraprendere, insieme al Parlamento, un percorso atto a verificare la situazione in Italia anche attraverso le associazioni che in questo senso operano nel territorio di valutare, insieme al Parlamento, la predisposizione di una legge precisa che vieti espressamente il matrimonio forzato, intervenendo in un'ottica di prevenzione anche su quanti rientrano da Paesi molto poveri in cui questa pratica è diffusa.

secondo le stime del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, 13,5 milioni di ragazze ogni anno nel mondo sono costrette a sposarsi in minore età; 37.000 bambine adolescenti ogni giorno sono costrette a matrimoni forzati. Ho sottoscritto la mozione n. 637 - e ringrazio molto la vice presidente Valeria Fedeli per averla promossa perché sono convinta che, di fronte a un fenomeno così grave come quello dei matrimoni precoci, abbiamo il dovere di impegnarci e di realizzare azioni concrete. Lo dobbiamo alle bambine e alle ragazze alle quali viene negata nei fatti l'infanzia; la negazione di un vissuto che comporta inevitabilmente la cancellazione della possibilità di una vita adulta autonoma, libera e autodeterminata. Fra le discriminazioni e le gravi violazioni dei diritti umani, cui è soggetto il genere femminile nel mondo, questa è senza ombra di dubbio la più grave e aberrante. L'imposizione del matrimonio, e la violenza sessuale ad esso correlata, a milioni di di bambine e adolescenti le espone infatti a lesioni fisiche e a gravi rischi per la salute, con danni irreversibili dovuti alle gravidanze e ai parti precoci e mette a repentaglio la loro stessa vita. Basti pensare che, secondo uno studio, le gestanti di età dai dieci ai quattordici anni hanno 5 volte più probabilità di morire durante la gravidanza o il parto rispetto alle donne di venti-ventiquattro anni. Senza contare poi che il matrimonio precoce coincide con l'abbandono scolastico e finisce per bloccare ogni potenzialità di sviluppo della persona. Le spose bambine sono spesso segnate da da depressione e suicidio per i gravi danni psichici che derivano dal vivere una condizione di vera e propria schiavitù sessuale. È solo del 2 luglio 2015 la prima risoluzione delle Nazioni Unite sulla prevenzione e l'eliminazione dei matrimoni forzati. La risoluzione, nel ribadire che i matrimoni precoci e forzati rappresentano una violazione dei diritti umani, si rivolge agli Stati e sottolinea l'importanza del coinvolgimento della società civile tutta per rafforzare il monitoraggio e gli interventi di prevenzione per contrastare questo fenomeno. La mozione n. 637 si muove nel solco di quella risoluzione, chiedendo quindi impegni molto precisi al nostro Governo. È importante e urgente che anche il nostro Paese si doti, a questo proposito, di una legislazione adeguata nel solco di quella svedese.

che riguarda prevalentemente i Paesi del Continente africano ed asiatico, ma che con l'aumento delle immigrazioni rischia di crescere anche in Europa e nel nostro Paese. Non abbiamo dati perché le indagini per quanto concerne le comunità di stranieri extracomunitari che in Unione europea negano i diritti delle bambine sono discontinue, ma è un fenomeno che richiede la nostra massima attenzione, così come quello delle infibulazioni genitali femminili. In queste settimane, in Commissione infanzia e adolescenza, è in corso un'indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori nell'ambito della quale presteremo la dovuta attenzione a questi temi. Ritengo inoltre, e concludo, che vada considerata l'importanza del ruolo della scuola. La scuola è fondamentale per realizzare una concreta integrazione. Per questo vanno promossi e incentivati progetti nell'ambito scolastico

rivolti alla prevenzione di questo fenomeno e alla promozione quindi di una cultura rispettosa dei diritti delle bambine e delle ragazze che bandisca definitivamente i matrimoni forzati. Mai più spose bambine; per raggiungere questo obiettivo, oggi quasi utopistico data l'enormità del fenomeno nel mondo, abbiamo il dovere morale, ancor più che politico, di agire in ambito internazionale e nel nostro Paese, difendendo i diritti, la dignità e la vita stessa delle bambine. Ne va della nostra stessa umanità.

nel quale abbiamo voluto proporre l'introduzione del reato di costrizione al matrimonio e di induzione al viaggio finalizzato al matrimonio di minorenni. Credo sia importante valutare la nostra proposta anche perché a me personalmente è risultato davvero sorprendente che l'Italia non si sia ancora dotata all'interno del proprio codice penale di questa fattispecie di reato,

Stiamo parlando di almeno 15 milioni di donne minorenni che, ogni anno, sono state costrette o si sono comunque sposate in età minorile.

di tutto il territorio e di ciò che accade all'interno dei luoghi di culto di altre religioni, in cui potrebbero essere celebrati matrimoni tra uomini e bambine. di un fenomeno di una gravità inusitata, perché un matrimonio precoce impedisce completamente ad una persona, ad un bambino di godere di diritti quale l'istruzione,

fino a due anni per chi induce al viaggio finalizzato al matrimonio. Quest'ultimo è un fenomeno grave e dobbiamo strutturare un'ipotesi di reato che deve risultare efficace e, soprattutto, applicabile. Ciò che accade in Italia - e vi sono moltissime testimonianze al riguardo - è che vi sono delle bambine che magari arrivano a confidare, fortunatamente, alla maestra o alla compagna di giochi

Per questa ragione speriamo che non ci si limiti solo a una mozione: dobbiamo infatti arrivare a un disegno di legge il più possibile condiviso per prevedere l'ipotesi di reato, perché anche il viaggio deve essere fermato

sarà però sufficiente, perché non basta una norma contenuta nel codice penale: occorre fare una grandissima campagna di sensibilizzazione perché queste bambine

Presidente, egregi colleghi, la mozione oggi in discussione richiama la nostra attenzione su un fenomeno di natura

casi come quelli che cerchiamo di rappresentare con i numeri di carattere globale che abbiamo citato. A me sembra, quindi, che l'iniziativa della collega Fedeli e delle altre college senatrici

che richiede l'intervento delle autorità scolastiche, degli insegnanti, dei servizi sanitari e sociali, dei pubblici ministeri e dei medici di famiglia, oltre che di quelli ospedalieri, per monitorare e combattere una prassi inaccettabile. Nessuno può chiamarsi fuori, nessuno può girarsi dall'altra parte o scegliere la strategia del silenzio, a proposito della quale propongo una ulteriore e conclusiva - per quanto riguarda il mio intervento - riflessione politica. La strategia del silenzio, purtroppo, è più estesa di quanto non appaia. È il frutto di una opzione culturale che dobbiamo abbandonare. È l'opzione in base alla quale c'è un malriposto senso di rispetto per culture diverse che non meritano di essere rispettate. Lo dobbiamo dire con molta franchezza e assertività:

non solo non vanno rispettate, magari proprio in nome della loro diversità, ma vanno apertamente contrastate e sanzionate. Un po' tutti siamo chiamati a questo compito, perché dobbiamo tutti stare in guardia nei confronti delle culture che propongono comportamenti inaccettabili dal punto di vista della tutela dei diritti umani e che, in quanto culture, in quanto prassi, a volte pretendono e riescono a diventare legge, anche se si tratta di leggi autodeterminate e illegittimamente determinate. Noi dobbiamo ribadire - lo deve fare il Parlamento in primo luogo - che nella Repubblica nessuno ha il diritto di proclamare la propria legge; che l'unica legge è quella della Repubblica e che la legge della Repubblica è la legge che risolve, in sé, ogni forma di legislazione e che nessun'altra forma di legislazione è tollerata nella Repubblica. Grazie, presidente

Su questo tema, infatti, non può esserci una discriminazione di interpretazione o di sensibilità. Questo è un tema che inerisce i fondamenti dei diritti umani, che, appunto essendo fondamentali, appartengono a tutti e ad ognuno. e ad ognuno. I dati sono certamente drammatici. Sono stati richiamati negli interventi che mi hanno preceduto. Ricordiamo che ogni sette secondi nel mondo una ragazza di meno di quindici anni si sposa, spesso con un uomo molto più grande di lei. A tutt'oggi abbiamo più di 700 milioni di donne sposate prima dei diciotto anni, delle quali un terzo sposate prima dei quindici

In ragione anche di una stima futura, si prevede che nel 2030 oltre 950 milioni di donne saranno sposate, e giovanissime. E nel 2050, addirittura oltre un miliardo e mezzo di giovani minorenni saranno costrette a matrimoni che (è importante richiamarne l'aggettivazione) saranno precoci e forzati.

può rappresentare un argomento ancillare, che va cioè a occupare un piano sottostante. A me così non sembra, perché quando un'Aula del Senato si confronta su queste tematiche,

Qualcuno ha detto che questi dati caratterizzano solamente alcune zone del mondo. A me non risulta, perché da un'indagine più approfondita, se è vero che nell'Africa subsahariana si contano approssimativamente (e per difetto) circa 39 milioni di matrimoni precoci e forzati,

che i diritti fondamentali che non vengono riconosciuti e che sono mortificati e offesi, non hanno solamente una collocazione di ordine religioso, ma diventano il portato di una cultura cui alcune figure si trovano ad assumere una posizione subordinata ad altre nell'assetto sociale. Credo che questo sia il tema che deve coinvolgere il Senato nei possibili provvedimenti che ne conseguiranno.

il Sottosegretario per gli affari esteri, che dà la dimostrazione di come evidentemente questo sia un tema che deve interessare anche la diplomazia e i contatti a livello internazionale. Infatti, è vero che la cultura viene affermata attraverso l'enunciazione di alcuni principi (Carta dei diritti fondamentali, Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), ma è anche vero che lo stesso Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite

Il passaggio che a me preme sottolineare però è il seguente: l'enunciazione di principi e il riconoscimento dei diritti sono sicuramente fondamentali, ma non possono essere esaustivi, perché i principi e i valori di riferimento non devono essere imposti con la forza, ma trasmessi attraverso una procedura di ordine diplomatico, culturale ed economico che fa sì che, attraverso lo sviluppo sociale, si possano trarre le giuste conseguenze. Si potrebbe immediatamente pensare che ci sia una disparità ovvia tra una dimensione di libertà declinata in alcune realtà del mondo e una libertà negata in altre realtà

un aspetto importante, perché il processo educativo e la dimensione culturale passano attraverso gli organi a livello internazionale, ma devono essere trasferiti e fatti propri attraverso un procedimento che richiede non solo diplomazia, ma anche giusti ma anche giusti contatti. Infatti, lentamente con il progresso e con l'evoluzione si dà luogo anche alla riduzione, se non alla scomparsa, di un fenomeno estremamente drammatico. Io credo che questo sia uno degli aspetti che maggiormente caratterizzano la trattazione di questo tema. Ho voluto sottoscrivere convintamente - come dicevo all'inizio del mio breve intervento - questa mozione, perché essa delinea dei punti ben precisi di un percorso che che il Parlamento stesso può portare a termine o che d'altra parte, attraverso altri tipi di provvedimenti, può consentire di conseguire un risultato tanto auspicato. Infatti in questa mozione si chiede al Governo di attivarsi, nelle sedi internazionali, al fine di garantire il pieno rispetto, da parte dei Paesi che ne sono firmatari, della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; ad assumere tutte le opportune iniziative per la piena attuazione della risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, alla luce della grave violazione dei diritti umani, oltre che di ogni principio di civiltà, che comporta il perpetrarsi della pratica dei matrimoni forzati; per ultimo, ma non ultimo, a valutare in uno scambio sinergico con il Parlamento l'opportunità di dotare l'Italia, in linea con l'esempio virtuoso della Svezia (già menzionata), di un'apposita normativa, al fine di configurare quale nuova fattispecie delittuosa il matrimonio forzato e tutte le attività connesse.

credo vada a sintetizzare nobilmente quello che ho cercato di trasmettere ai colleghi: che sia l'ultima volta - così dice Malala - che un bambino o una bambina spendono la loro infanzia in una fabbrica, che sia l'ultima volta che una bambina sia costretta a sposarsi e che sia l'ultima volta che un bambino innocente muoia in guerra. Che vuol dire questo? Vuol dire che ciò di cui stiamo trattando oggi è un aspetto,

Signor Presidente, anch'io ringrazio la nostra Vice Presidente e mi sento anch'io coprotagonista in questo percorso. cominciare dalle parole che ha appena pronunciato il senatore Romano, perché purtroppo, nonostante la profonda condivisione, la convinzione e il riconoscimento che il mondo ha fatto alla giovane Malala, il suo auspicio ancora oggi e ancora in questo momento viene tradito. Ed è tradito perché abbiamo detto e ripetuto dati che non sono numeri: ogni sette secondi, quindi già durante questo nostro confronto, quante bambine sono state date in spose?

queste bambine sono date in spose sono sconosciuti che le comprano come cose al mercato, che le useranno come schiave, che abuseranno di loro, che le priveranno della possibilità di studiare e di frequentare coetanei, che le obbligheranno ad avere gravidanze precoci e indesiderate, con conseguenze gravissime, a volte mortali. Il circolo vizioso che riguarda i matrimoni infantili racchiude in sé, quindi, una miscela di fattori davvero nefasti: alta possibilità di abbandono scolastico, possibilità di contrarre malattie veneree davvero terribili, come l'HIV, che in quei Paesi non vede ancora riconosciuto il diritto alle cure, o di morire a causa di complicazioni durante la gravidanza o il parto. Sappiamo bene, infatti, che la seconda causa di morte per le ragazze, dopo i suicidi, è rappresentata proprio dalle gravidanze e dal parto. E tutto questo ha una paternità e una maternità bei definiti: guerra, povertà, discriminazione di genere, mancato accesso all'istruzione. A volte, sono le stesse famiglie che, pur di dare una speranza di vita alla propria figlia, la cedono come fosse un oggetto, trattandola al pari di una cosa. Vediamo quanta disperazione c'è in questo gesto. Tutto questo è inoltre inesorabilmente amplificato e diventa particolarmente evidente in momenti tragici e di guerra, come quelli che stanno ora vivendo alcuni Paesi nel mondo, come la Libia o la Siria, dove tale pratica, a volte, rappresenta l'unico modo per salvare una ragazza da ulteriori nefandezze, come stupri o violenze, che aumentano purtroppo vertiginosamente nei casi di conflitti armati lunghi e cruenti. Sappiamo anche come in certi Paesi, in Africa ad esempio, alcuni genitori, privi di ogni possibilità di reazione (non possono neanche difendersi), sono costretti a subire veri e propri rapimenti dei propri cari, a subire un destino che certamente non vorrebbero. Mancanza dei minimi livelli di istruzione, povertà e presenza di culture che spesso relegano le donne in fondo alla piramide sociale contribuiscono a creare quella fragilità di cui le bambine, poi, rimangono vittime.

Tornando al problema delle spose bambine, dobbiamo rilevare come anche nel nostro Paese, con l'aumento dell'immigrazione di persone provenienti dal subcontinente indiano e dai Paesi arabi, portatrici di culture molto differenti dalla nostra, sia aumentato il fenomeno dei matrimoni forzati. Con la presenza delle seconde generazioni il matrimonio, da combinato, è diventato forzato. Questo implica un processo di violenza psicofisica, quasi sempre misconosciuto, del quale prendiamo coscienza e consapevolezza soltanto quando si verifica un fatto di cronaca eclatante, come abbiamo visto. non è ineludibile, si può e si deve cambiare. Infatti, le scelte politiche dei Governi nazionali possono cambiare le cose nel mondo: la prima inderogabile opzione parte dall'esigenza di creare un'istruzione adeguata e livelli minimi indispensabili. Lasciatemi Lasciatemi aggiungere solo che cultura e istruzione rappresentano i due pilastri da cui partire per poter cambiare la vita di interi popoli e Nazioni e per contribuire a realizzare un mondo più giusto, senza il quale non ci può essere pace. Solo l'accesso all'istruzione per tutte quelle bambine attualmente escluse potrà davvero salvare il mondo.

quali viene letteralmente tolta l'infanzia e che spesso sono sottoposte a soprusi e a violenze. Oltre all'aggravante di doversi sposare con persone a loro non gradite, in un'età molto fragile, subiscono violenze di tipo fisico e psicologico. Il fenomeno non è connesso solo alla guerra e alla povertà, ma spesso anche all'ignoranza ed è sostenuto da leggi antiche, quasi tribali, che, in assenza di un livello culturale appropriato, vengono semplicemente accettate e imposte a queste ragazze, non hanno alcun potere di scelta, sono isolate dalla società civile e private dell'infanzia. Questo è l'aspetto peggiore perché ovviamente viene tolta loro la libertà e la possibilità di autodeterminarsi.

del denaro da chi la prende in moglie. I numeri di questa pratica sono allarmanti. Vengono citati anche da un articolo de «l'Espresso»

Ci sono casi di ragazze giovanissime, appartenenti a famiglie di immigrati ma italiane, anche da un paio di generazioni, forzate a tornare al Paese di origine per essere date in spose. Siano chiari due punti: in primo luogo si tratta di ragazze italiane che è dovere dello Stato proteggere e tutelare. Sono italiane nei fatti perché spesso queste ragazze vivono qui, sono immigrate di seconda generazione, ma non hanno la cittadinanza. Forse quindi sarebbe il caso

che si trova in un altro Paese. La nostra civiltà deve essere migliore di così, più forte delle usanze e credenze popolari e certamente deve scoraggiare qualsiasi atteggiamento di disinteresse che si mascheri dietro il ridicolo commento: sono straniere. Queste ragazze non solo perdono la loro infanzia, e contestualmente la loro felicità, per sempre, ma spesso rischiano la vita a causa delle violenze e dell'esperienza traumatica

partire dal nostro territorio per far sì che vi sia una migliore istruzione anche per le persone che vivono in un ambito familiare e in un contesto culturale e religioso diverso dal nostro.

donne molto piccole. Credo, quindi, sia importante un'educazione sentimentale nel rispetto delle parti, e questo lavoro va fatto insieme agli uomini proprio per creare un rispetto dei sentimenti e fare in modo che queste cose non avvengano.

la mozione della senatrice Fedeli, di cui sono cofirmataria e alla quale mi riferisco, intende impegnare il Governo su tre punti rispetto al fenomeno delle spose bambine, i cui dati sono stati riportati dalle cronache ieri, in seguito al *report* diffuso martedì da Save the Children, in occasione della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Le statistiche portano alla nostra attenzione dati medi molto preoccupanti, ma i dati singoli, troppo frequentemente, sono spaventosi: bambine date in sposa addirittura a sei/otto anni, costrette a rapporti sessuali la notte stessa del matrimonio, forzate da un marito che né conoscono né tantomeno hanno liberamente scelto, a dispetto delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e degli accordi stipulati tra le famiglie.

I problemi però non riguardano solo i matrimoni e le maternità precoci, che, per via della struttura fisica ancora da sviluppare e della condizione fisiologica immatura delle madri bambine, comportano enormi rischi per la loro salute e per la vita loro e dei loro figli. L'Unicef ha diffuso dati secondo cui le bambine tra i cinque e i quattordici anni sono occupate il 40 per cento in più del tempo (circa 160 milioni di ore in più al giorno), rispetto ai ragazzi della stessa fascia di età, in lavori domestici non pagati nonché nella raccolta di acqua e di legna. Si stima che le ragazze tra i dieci e i quattordici anni in Asia meridionale, Medio Oriente e Nord Africa sono occupate circa il doppio del tempo in faccende domestiche rispetto ai ragazzi, e che solo una femmina ogni tre maschi frequenta la scuola secondaria. L'Agenzia ONU ipotizza che un miglioramento di questo dato del 10 per cento alzerebbe il PIL del 3 per cento, ma questo argomento non vale, niente da fare; all'interno di una situazione desolante per l'infanzia nei Paesi poveri - secondo un rapporto Unicef-Banca mondiale, 385 milioni di bambini vivono in povertà estrema - quella delle bambine rappresenta una posizione doppiamente perdente. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché voglio rivolgere con forza un appello al Governo affinché si impegni nel senso di questa mozione, ma vorrei anche cogliere l'occasione per riportare l'attenzione delle onorevoli colleghe e colleghi alla mozione che abbiamo discusso ieri in quest'Assemblea e con cui si impegna il Governo nella lotta all'obesità. Lo faccio per rilevare che nel giro di due giorni ci siamo occupati, da un lato, dei sintomi e degli effetti di una civiltà che si perde nella spirale di risorse sprecate; risorse sprecate per riempire con cibo spazzatura il vuoto del non senso della propria esistenza, per promuovere campagne in favore di stili di vita e di alimentazione sani, per curare le patologie legate all'obesità: quanti soldi spesi in lassativi, in antidepressivi, in chirurgia estetica, in palestra, in benessere, in *junk food* ! E non estendo il ragionamento. Dall'altro lato, oggi ci occupiamo degli effetti di una civiltà che si cancella nella spirale della povertà, perché ricordiamo che quello delle spose bambine è un fenomeno in larga parte legato alla povertà, la quale accentua, giocoforza, le criticità legate alla loro cultura e alla loro religione; una civiltà che si cancella nella spirale della fame,

La politica si deve attivare affinché a livello internazionale, come nel nostro Paese, ci si doti di strumenti di programmazione e di contrasto, ma sarà sempre un lavoro fatto soltanto a metà, se queste discussioni e questi impegni non sono anche un'occasione per mettere in luce le nostre dirette responsabilità rispetto alla condizione di estrema povertà in quei Paesi.

anche e soprattutto quella recente, e in cui non dobbiamo perdere l'opportunità di riflettere in modo critico sui nostri modelli di consumo, sulle nostre soluzioni alla crisi attuale, sulla nostra condizione di vita, sui nostri privilegi, privilegi, che talvolta tramutiamo in diritti che, se visti in chiave storica e sistemica, sono in realtà indifendibili nonché in netta contraddizione con le nostre varie posizioni. Il tempo a mia disposizione non mi permette di affrontare i ragionamenti ai quali ho genericamente accennato in chiusura, ma non dimentichiamoci di illuminare anche questa visuale. Signor Presidente, voglio iniziare raccontandovi una storia, quella di Rubina, di 400 euro e di una bicicletta. Rubina era una bambina come tante; il suo unico problema era quello di essere nata in uno Stato, il Bangladesh, dove la sua dignità di minore era calpestata quotidianamente. Ormai da qualche anno, infatti, Rubina, nel pieno del suo sbocciare, veniva molestata da uomini e ragazzi del suo villaggio. La famiglia, allora, decise di farle un regalo il giorno del suo dodicesimo compleanno: per contrastare le molestie che subiva quotidianamente nel suo villaggio e per non infangare il nome della discendenza, si decise che era arrivato il momento di darla in moglie. Nessuno chiese alla piccola Rubina la sua opinione e nessuno si domandò quale fosse il suo volere. Così Rubina, da poco dodicenne, fu costretta a contrarre matrimonio dando l'addio per sempre alla propria infanzia, portando in dote 400 euro e una bicicletta. Rubina era una bimba come tante, andava a scuola e giocava con le amiche. Fu proprio la scuola, e in particolare un professore, a volerla riportare sui banchi della sua classe. E grazie a questo intervento i genitori decisero di rinviare le precoci nozze. Ma, come ogni brutta storia, arriva un epilogo spiacevole. La piccola risultava sempre più assente alle lezioni; assenza che la famiglia mascherava con malattie e scuse banali. Allora, il buon maestro bussò per l'ennesima volta a casa di Rubina per chiedere spiegazioni, ma gli fu detto che si trovava dai nonni a festeggiare la fine del Ramadan. Tornato a scuola, sconfortato, i compagni di scuola gli raccontarono una agghiacciante verità: la bambina si era sposata e ormai viveva con il marito, un uomo adulto molto più grande di lei. A questo punto il professore tornò a casa della piccola Rubina e cercò di avere conferme: dopo diverse insistenze, la madre ammise il matrimonio della figlia. Un mese dopo, Rubina scelse di morire. Il suicidio di Rubina si può ritenere una sconfitta per tutti. Una sconfitta per la famiglia che cercava di proteggerla e che l'ha costretta, ad appena dodici anni, a sposarsi con un uomo molto più grande di lei,

per quel professore testardo e per la scuola intera, che non è riuscita a salvare la bambina, nonostante i progetti contro l'abbandono. Una sconfitta per le associazioni come Terre des Hommes che portano avanti campagne di informazione sulla tratta delle spose bambine che finiscono nei bordelli delle città, oppure sfruttate nelle fabbriche della capitale. Ma soprattutto, la morte di Rubina è una sconfitta per tutti, tutti quelli che oggi hanno la possibilità di fare qualcosa e che si girano dall'altra parte. «Abbiamo cercato di aiutarla senza riuscirci» - dicono i volontari dell'associazione Terre des Hommes - «ma questo rafforza ancora di più la nostra convinzione che le sue compagne, e le ragazzine di tutto il mondo, abbiano più che mai bisogno di essere protette, sostenute e aiutate a diventare le protagoniste del futuro». Allora noi, in quest'Assemblea, possiamo finalmente adoperarci per tutte quelle bambine come Rubina, che pur di scappare da situazioni disumane preferiscono percorrere la via del suicidio. Vale la pena ribadire cosa possiamo fare e cosa può fare oggi questo Governo affinché nessuno possa raccontare di nuovo la storia di Rubina o di un'altra come lei. Cosa chiediamo? Chiediamo all'Esecutivo di attivarsi, mediante l'utilizzo di ogni utile mezzo, presso le competenti sedi nazionali e internazionali, affinché siano compiuti tangibili passi volti al contrasto del fenomeno delle spose bambine, della violenza di genere contro le donne e dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i generi, soprattutto in via preventiva, mediante l'adozione di politiche efficaci e di concrete misure da attuarsi specie nei territori maggiormente a rischio, dando seguito ai precetti contenuti nella Convenzione di Istanbul e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Questo è un importante passo, perche è assurdo che nell'attuale contesto sociale e culturale a livello globale si debbano ancora piangere queste morti. fondamentale assumere ogni necessaria azione affinché si proceda in tempi brevi a una compiuta raccolta, da parte degli organismi istituzionali, degli enti e delle organizzazioni competenti, dei dati inerenti al fenomeno delle spose bambine, nonché al successivo monitoraggio, studio e controllo, per ostacolare fattivamente tale ripetuta violazione dei diritti umani. Solo con le carte in mano saremo in grado di comprendere la portata reale del fenomeno, finora oscuro. È necessario incentivare, anche attraverso il coinvolgimento attivo delle organizzazioni internazionali governative e non governative riconosciute, un efficace piano di educazione ai diritti per le fasce di età maggiormente esposte, per il rafforzamento della coscienza civica, a partire dall'età scolare, dell'autonomia e dell'autodeterminazione delle donne anche in tema di salute sessuale e riproduttiva. Questi punti sono fondamentali per il raggiungimento della parità di genere. altrettanto importante adoperarsi affinché, a partire dal contesto nazionale, ove si riscontri un vuoto precettistico, ogni Paese attualmente inoperoso implementi in maniera puntuale e cogente il proprio quadro normativo, mediante la previsione di specifiche fattispecie delittuose, sufficientemente sanzionatorie, sul matrimonio forzato. In ogni Nazione dobbiamo finalmente scrivere a caratteri cubitali la parola fine a questa abominevole pratica, che deve trovare un arresto con condanne certe. Bisogna garantire e promuovere, anche negli idonei ambiti extraterritoriali, un'apposita protezione e la garanzia dell'anonimato per tutte le bambine e le ragazze che intendano denunciare reati e minacce, anche mediante uno specifico impegno di ricezione e opportuna trasmissione da parte degli operatori sanitari. operatori sanitari. L'omertà è infatti uno dei fattori che maggiormente ostacola l'emersione del fenomeno e della realtà. Le piccole donne del domani, acerbe spose di oggi, devono essere messe nella condizione di raccontare gli abusi e sentirsi protette. In ultimo, bisogna sostenere, anche nel contesto del dialogo e del confronto tra le Nazioni in tema sanitario e di tutela dei diritti, nel caso di pericolo di vita della madre minorenne esposta a violenze e coercizioni e del feto, alla presenza di condizioni igienico-sanitarie adeguate, il riconoscimento della pratica dell'interruzione di gravidanza, nonché un idoneo successivo percorso di assistenza psicosociale. Il corpo di queste bambine non può sostenere il peso di una simile violazione fisica e morale, in quanto esse ne escono sfigurate, con cicatrici che si imprimono davvero nel corpo e che rimangono per sempre nell'anima.

Solo così, un briciolo di giustizia sarà fatto anche a nome di Rubina.

che non so quanto recepiranno della nostra discussione. Nei Parlamenti le discussioni politiche sono anche rivolte a tutelare grandi principi, al di là delle

fondante delle convenzioni internazionali nonché di leggi nazionali, ma che purtroppo è spesso contraddetto nella realtà quotidiana da atteggiamenti culturali e politici adultocentrici; quegli atteggiamenti che piegano il diritto superiore del bambino ai propri desiderata, alle proprie personali convenienze e opinioni. La piaga dei matrimoni precoci è uno dei tanti diritti negati all'infanzia. Basti pensare al tema dei bambini soldato, al lavoro minorile, ai maltrattamenti, agli abusi, alla prostituzione minorile. Ma all'interno di diritti negati ai minori, i diritti delle bambine sono ancora più calpestati e la piaga dei matrimoni precoci è esattamente uno di questi diritti negati. Si tratta di una terribile violazione dei diritti umani delle bambine; bambine a cui viene rubata la vita. Si tratta di un furto di vita, perché viene negata loro la possibilità di sognare e progettare la propria vita, nonché di progredire, di migliorare il proprio futuro e di essere padrone del proprio destino. destino. Il matrimonio precoce blocca infatti il loro percorso scolastico e d'istruzione e compromette la loro salute psicofisica. Ricordo che ogni anno 70.000 bambine muoiono per cause legate al parto e alla gravidanza. Voglio ricordare che gran parte dei Paesi in cui è massicciamente praticato il matrimonio precoce, sono anche Paesi in cui è elevatissimo il ricorso all'infibulazione, con tutte le conseguenze psico-fisiche e sanitarie che questo comporta. Le conseguenze del matrimonio precoce riguardano naturalmente le bambine che lo subiscono, ma vanno oltre la loro vita di spose bambine perché colpiscono anche le generazioni successive alla loro. loro. Le spose bambine sono infatti costrette ad abbandonare la scuola e questo limita non solo la loro personale prospettiva futura, ma anche la loro abilità e possibilità di crescere figli in modo libero, di contribuire alla crescita sociale ed economica propria e dei propri figli. I figli di una madre bambina non alfabetizzata, infatti, non avranno a loro volta un facile ingresso a scuola o, peggio, le figlie di una sposa bambina analfabeta molto più facilmente abbandoneranno la scuola, si sposeranno giovani e inizieranno di nuovo quel circolo vizioso della povertà e della negazione fondamentale di diritti umani. Noi, anche con questa mozione e con gli atti che ne conseguiranno, vogliamo spezzare questo circolo vizioso, restituendo alle bambine il loro diritto ad essere tali, il loro diritto a scegliere chi amare e quando amare quando sarà l'ora, il loro diritto a crescere diventando donne libere ed autonome. La comunità internazionale, come ricordava un altro collega, si è impegnata a mettere fine ai matrimoni precoci entro il 2030. Se però il *trend* rimarrà quello attuale, nel 2030 avremo 950 milioni di spose bambine; 250 milioni in più dell'attuale dato. Ciò che serve è una serie di azioni, ma in primo luogo una battaglia di carattere culturale nel mondo, ma anche in Italia. Anche in Italia dobbiamo aprire gli occhi, non chiuderli, dobbiamo esplorare e monitorare bene la realtà. Quella realtà che ci descrive ci descrive il lavoro di molte associazioni, che ci dice che anche in Italia, a causa dell'incremento dell'immigrazione delle famiglie provenienti dal subcontinente asiatico e da alcuni ai Paesi arabi, si è sviluppato ed è aumentato il fenomeno dei matrimoni forzati. È davvero importante questa mozione, che impegna il Governo ad attivarsi nelle sedi internazionali anche per garantire il pieno rispetto delle Convenzioni sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché a dotare l'Italia, in analogia alle scelte della Svezia, di una normativa che configuri il matrimonio forzato e tutte le attività connesse quale nuova fattispecie delittuosa. Accanto a questo serve però una responsabilità collettiva, di tutte le istituzioni e della società civile. Dico ciò rispondendo anche alle preoccupazioni che esprimeva poco fa il senatore

Grazie,

parole da «a garantire» fino a «professione medica», sostituendole con il seguente paragrafo: «a rafforzare e potenziare gli strumenti di tutela sia preventivi che repressivi dei diritti delle vittime dei reati in oggetto, valutando anche eventuali modalità di coinvolgimento e impegno degli appartenenti alla professione medica». alla professione medica; 6) a sostenere, in armonia con le disposizioni nazionali, anche nel contesto del dialogo e del confronto tra le nazioni in tema sanitario e di tutela dei diritti, nel caso di pericolo di vita della madre minorenne esposta a violenze e coercizioni e del feto,

Grazie,

di alcune bambine in particolare, ma sono poche delle quali siamo venuti a conoscenza. Penso a Rubina, la bimba che si è impiccata nella casa di quegli stessi genitori che l'avevano donata stata costretta a sposare; o al caso ancora più drammatico di Rawan, morta a soli otto anni durante la sua prima notte di nozze, il cui decesso è stato causato dall'emorragia dovuta alle lesioni provocate dal rapporto sessuale con il marito quarantenne. I numeri che ci richiamano a una drammatica realtà sono quelli per cui ogni sette secondi una ragazza con meno di quindici anni si sposa;

Detengono il triste *record* i Paesi più poveri: da quelli africani all'India, che detiene il ben poco invidiabile primato del più alto numero in assoluto, con il 47 per cento delle ragazze

numeri drammatici, che non possono passare sotto silenzio. Le mozioni oggi in esame riguardano proprio uno dei drammi della nostra epoca, un dramma che colpisce sicuramente aree geografiche del mondo dove sottosviluppo, ignoranza, pregiudizi (talora anche di carattere religioso) orientano verso determinati tipi di scelte, ma è un problema che purtroppo arriva ad interessare anche Paesi come il nostro con il diffondersi dei fenomeni migratori. Le conseguenze per queste bambine sono tremende dal punto di vista innanzitutto della scolarizzazione, con la fine di ogni progetto di istruzione e con essa di ogni reale possibilità di uscire da una condizione di sudditanza, di dipendenza; in pratica, è la prospettiva per queste ragazze di restare quasi schiave a vita, senza poter neanche sognare una soluzione diversa per il proprio avvenire. Per non parlare poi delle conseguenze di carattere sanitario e psicologico, che non sono meno tremende, perché anche laddove non si ricorre all'aborto, la gravidanza in età così precoce costituisce un rischio maggiore dal punto di vista della salute per il bimbo che nascerà, oltre che per la sua mamma. Cosa fare? Le mozioni ci invitano ad agire. Dobbiamo impegnarci in quei Paesi in cui questa pratica è occulta, in quelli dove è diffusa, compresi quelli che hanno stabilito per legge l'età minima per il matrimonio, l'istruzione obbligatoria si trovano di fronte ad una realtà in cui le norme tradizionali di ordine culturale continuano ad avere il sopravvento sulle buone leggi approvate. Sono fondamentali la prevenzione, la scuola, il sistema educativo, nel quale è più elevata la probabilità di entrare in contatto con minorenni e giovanissime destinate al matrimonio contro la loro volontà. Si tratta Si tratta di interventi complessi, non semplici, che mettono in gioco legami affettivi con la famiglia, si muovono in un terreno difficile, scivoloso, tra attaccamento e rifiuto della tradizione, in quella frontiera del confronto tra identità originarie e modernità della cultura occidentale. La scuola potrà essere anche luogo in cui avviene la formazione di una coscienza dei diritti, che valorizzi sin da piccole il valore della libera scelta di vita delle donne, in cui anche le famiglie stesse si possano aprire in un dialogo, praticare lo scambio, la contaminazione:

ma ciò che occorre sono anche le condizioni materiali adeguate a garantire la protezione, laddove ci può essere una denuncia o una ribellione. Insomma, sono i principi della società che devono cambiare, perché è vero che quando si pratica la barbarie si diventa barbari, ma è anche vero che chi tollera la barbarie nel silenzio si fa barbaro. Ci aspettano allora, ancora una volta un cammino di civiltà tanto impegno, quello che la nostra stessa storia ci impone, per affrontare, nel fenomeno dell'immigrazione che il nostro Paese subisce, anche questo. questo. La questione dell'immigrazione ha infatti posto all'attenzione del nostro Paese pratiche drammatiche che avvengono nel silenzio delle nostre città, quella dell'infibulazione. Molte comunità, infatti, autotutelandosi, proteggendosi e impedendo alle nostre forze sociali - a quelle sentinelle sul territorio che siamo noi, le forze di polizia e di sicurezza e molte altre istituzioni, scuola compresa - e ai nostri occhi di vedere e alle nostre orecchie di sentire, perpetuano nel nostre Paese le loro tradizioni e la loro cosiddetta civiltà. E noi nel confronto tra civiltà, nell'ospitare queste persone e il grande fenomeno dell'immigrazione, ci interroghiamo su cosa sia davvero l'integrazione e se noi per integrazione intendiamo per caso - spero di no

quale per prima ha posto all'attenzione di quest'Aula un tema che a noi sembra così lontano ma che, in realtà, è così vicino. non segna la presunzione di voler modificare la cultura e le tradizioni altrui, ma segna, invece, la grande ambizione di vedere i diritti fondamentali e basilari di ogni donna e di ogni età, tutelati e garantiti in tutti i Paesi, a partire dal nostro. a partire dal nostro. Il dibattito di stamane, prezioso per i contributi giunti da uomini e donne, che nel loro mandato parlamentare guardano con attenzione all'umanità dolente che questa pratica racconta, sia l'inizio di un percorso legislativo molto rapido, perché il nostro Paese non sia tra i Paesi indifferenti e si doti presto - prestissimo - di una legge che sancisca che nel nostro Paese ogni ogni violenza contro le donne, di qualsiasi tipo e da chiunque provenga, è severamente vietata e punita dalla legge. Grazie, presidente Fedeli, e grazie alle colleghe che hanno ulteriormente arricchito con la presentazione delle loro mozioni questo dibattito. Grazie soprattutto ai colleghi uomini che sono intervenuti in questo dibattito,

alla mozione presentata dalla vice presidente Fedeli e, ovviamente anche alle altre mozioni presentate casomai non dovessero convergere in una unica sintesi, che anche io auspico, ringrazio soprattutto la Presidenza del Senato, che ha voluto così tempestivamente calendarizzare questa discussione.

è veramente sorprendente che nel 2016 ci si avveda che nel codice penale non è previsto un reato come quello dell'induzione al matrimonio di un minorenne o l'induzione a un viaggio finalizzato al matrimonio. Sembra quasi un atto di inciviltà o, forse, per anni si è pensato che il fenomeno potesse interessare soltanto Paesi stranieri, che abbiamo citato prima: Niger, Ciad, Bangladesh. Purtroppo, invece, il fenomeno si è intensificato. È un fenomeno che, sicuramente, non può non essere correlato all'immigrazione: un'immigrazione e una migrazione che hanno portato quasi interi popoli a spostarsi da un'area all'altra del mondo, arrivando in un territorio come quello italiano dove si rischia che non vi sia neanche il controllo del medesimo. Quando non vi è un controllo del territorio, non vi è il controllo di quello che accade all'interno dello stesso, perché probabilmente, se ci si domanda se qualche bambina in Italia possa andare in sposa

il compito di cui si deve fare carico tutta la comunità internazionale è quello di istruire le persone, perché solo la cultura e l'istruzione,

dobbiamo arrivare a un disegno di legge, il più possibile condiviso, per la previsione di tali reati in Italia. Accanto a ciò deve essere prevista una campagna di sensibilizzazione.

colleghi, un figlio, un bambino non denuncia il padre o la madre; occorrerà che la maestra, la professoressa, la compagna di scuola o i genitori della compagna di scuola diano un supporto alla bambina o al bambino che sono costretti

Dobbiamo combattere le cause che portano a questi episodi; dobbiamo combattere quel tipo di cultura e tradizioni, che all'origine ha portato a credere che bambini e bambine possano anche arrivare alle nozze,

ma che ebbe cura di consumare il matrimonio quando aveva nove anni; e questo è scritto su un testo di natura religiosa.

ma siamo noi che dovremmo insegnare quella cultura e quella civiltà che abbiamo la fortuna di avere attualmente. Per cui tutto il Gruppo della Lega Nord voterà a favore

i senatori e le senatrici di Sinistra Italiana voteranno con convinzione la mozione a prima firma della vice presidente Fedeli e quella a prima firma della senatrice Donno. Come Senato, abbiamo ritenuto assolutamente opportuni la discussione e il dibattito svolti, a distanza di pochissimi giorni dalla Giornata internazionale delle bambine

che fanno tremare e fanno dire ancora una volta che forse purtroppo nascere donna, nascere femmina, è ancora una disgrazia. Si tratta di dati che noi spesso ignoriamo e che non che non riguardano, come qualcuno vuol far credere, magari soltanto altri Paesi. Conosciamo perfettamente i dati della Nigeria, dell'Etiopia e dell'Asia.

stipulato un accordo vergognoso per il trattenimento dei migranti. Voglio leggere i dati che riguardano la Turchia. Stiamo parlando di 181.000 spose bambine ogni anno

queste mozioni, pensare di esserci lavati la coscienza, dicendo: «Oggi abbiamo fatto la nostra opera buona»;

Il fenomeno colpisce bambine e ragazze nei loro diritti fondamentali, alla salute e all'istruzione, impedendo loro di vivere l'infanzia, di realizzare i sogni e i progetti. A tutto questo si accompagna l'abbandono della scuola. Sono costrette a subire violenze domestiche, abusi, stupri, incorrendo in gravidanze precoci. Risultano particolarmente esposte alle malattie sessualmente trasmissibili, come l'HIV. Oltre tutto, le barriere amministrative e legali e le pratiche socioculturali e religiose in moltissimi Paesi impediscono a molte bambine e ragazze di accedere ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, come i *test* dell'HIV e i metodi contraccettivi.

La guerra è un elemento che peggiora in modo significativo le condizioni delle bambine e delle ragazze. Gli ultimi dati dell'ONU dimostrano che cento delle ragazze siriane tra i dodici e i diciassette anni rifugiate in Libano è stato costretto ad un matrimonio precoce; e questo è un altro dramma nel dramma della guerra. Ma dietro ogni cifra, ogni dato, vi è un volto, una storia. Hanno fatto bene molte Grazie, «Se non fosse stato per la guerra non mi sarei mai sposata così giovane. La guerra ha distrutto la mia vita e quella di tutti i siriani», dice Afrah, una *baby* sposa, fuggita da Al Rastan, città della Siria dell'Ovest, roccaforte dei ribelli, e rifugiata

più emarginati e vulnerabili della società: quasi sempre appartengono alle classi più povere. Per

per garantire il pieno rispetto, da parte dei Paesi che ne sono firmatari, della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, non solo assumere tutte le iniziative per la piena attuazione della risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite

e sappiamo che sarà un percorso lungo e complesso - richiedono una grande battaglia per l'informazione e la sensibilizzazione che consenta a tutte le donne, anche alle bambine, di conoscere i propri diritti. Serve una grande battaglia per l'istruzione, perché solo attraverso una forte capacità di garantire l'accesso alla scuola e all'istruzione potremo dare a queste bambine una nuova consapevolezza e anche gli strumenti per la loro liberazione e per combattere contro tutti i pregiudizi, per fare in modo che nel mondo non sia più una disgrazia, come i dati ci dicono, nascere donna.

Grazie, presidente nel mondo risultano esserci 700 milioni di donne che si sono sposate prima dei diciotto anni, e di queste il 17 per cento - 125 milioni - vive in Africa; una su tre di queste giovanissime donne africane si è sposata prima dei quindici anni. In Mauritania, il 60 per cento delle adolescenti ha un marito di almeno dieci anni più vecchio. Nella sola Nigeria le spose bambine sono 23 milioni. Bene, finalmente in quest'Aula oggi è stato attenzionato Il fenomeno si sta rivelando in tutta la sua gravità nel presente e ne abbiamo preso atto oggi in tutta la discussione e nelle illustrazioni delle mozioni. In futuro si rischia di raggiungere dati ancora più allarmanti, visto il legame sempre più stretto che si sta manifestando tra questo vergognoso fenomeno e le fasce più povere della popolazione,

se non si metteranno in atto le misure adeguate richieste dalle mozioni, nel 2030 avremo 950 milioni di donne sposate giovanissime. Questi sono i dati dell'indagine di Save the Children. È importante che si faccia una riflessione sul fatto che le guerre e le crisi umanitarie alimentano questo fenomeno. Anche noi ringraziamo la collega senatrice Fedeli per aver presentato una mozione che mette in luce la necessità di iniziative di contrasto ai matrimoni forzati

alle bambine più povere e marginalizzate, promuovendo interventi di prevenzione indirizzati soprattutto a un'istruzione di qualità, cosa che purtroppo, nel nostro Paese, non risulta

occasioni e opportunità per dare ai ragazzi maggiore consapevolezza dei diritti umani e dei propri diritti, purtroppo, come abbiamo visto,

compresa quella del nostro Paese. Ogni sposa bambina rappresenta una tragedia individuale; abbiamo ascoltato anche dalla nostra collega Donno una Donno una dimostrazione di ciò che accade, ma è solo un esempio. L'Italia purtroppo fino ad ora non ha profuso un grande impegno affinché si accendessero i riflettori su questa situazione. Per tale ragione, alla luce di queste brevi considerazioni, chiediamo al Governo impegni precisi affinché si avvii una complessiva e rigorosa raccolta dei dati (e ci sia realmente una raccolta dei dati inerenti al fenomeno delle spose bambine) si attivino al più presto il monitoraggio e lo studio richiesto nella mozione volto a contrastare la ripetuta violazione dei diritti umani. Chiediamo una serie di efficaci politiche di prevenzione, ispirate ai precetti contenuti nella Convenzione di Istanbul e in quella delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, da attuare nei territori maggiormente a rischio, soprattutto con l'incentivazione di un piano di educazione ai diritti per le fasce di età maggiormente esposte, per un rafforzamento della coscienza civica, a partire dall'età scolare, dell'autonomia, dell'autodeterminazione delle donne anche in tema di salute sessuale e riproduttiva, e anche per il

un'apposita normativa, prevedendo il reato *ad hoc* per chi induce o costringe a contrarre matrimonio. In Italia questo serve. Il dibattito è stato ricco e proficuo in questa Aula e ci ha fatto piacere anche rilevare la disponibilità del Governo nell'accogliere gli impegni.

È inerente a quanto stiamo trattando quest'oggi; è veramente allucinante quello che si legge. Mi riferisco ad un annuncio su eBay, di una neonata in vendita a 5.000 euro.

non può essere dimenticato, ma soprattutto non può essere sottovalutato. Aggiungo solo un dato per porre all'Assemblea una riflessione che - secondo me - dovremmo riprendere con prossime iniziative legislative. Noi non possiamo ignorare che nel mondo, ogni sette secondi, una bambina sotto i quindici anni viene data in sposa in modo forzoso in matrimonio precoce, e che più di un milione di bambine sotto i quindici anni subiscono delle gravidanze altrettanto forzose. Questi sono dati oggettivi. Va dato merito oggi alla senatrice Fedeli, e naturalmente a tutti noi, da lei sollecitati, di avere puntato i riflettori sul tema, ma sarebbero riflettori assolutamente inutili se non si desse un seguito legislativo a ciò di cui oggi stiamo parlando. Personalmente non sono favorevole, non lo sono mai stata, alla pan-penalizzazione selettiva, ossia all'identificazione di micro reati per ciascuna fattispecie. Esiste un codice penale, esistono fattispecie di carattere generale che possono coprire la più parte delle fattispecie delittuose. Ma in questo specifico caso abbiamo degli esempi significativi: li abbiamo nei Paesi nordici, come la Svezia, che citava giustamente la vice presidente Fedeli, ma li abbiamo anche in Germania, dove esiste il reato penale di matrimonio precoce e forzoso. Consegnando tutte le considerazioni, che sono state peraltro espresse in maniera eccellente dalle colleghe e dai colleghi che sono intervenuti in discussione generale e in fase di dichiarazioni di voto, vorrei però invitare tutti

sono bambine a cui sono sottratti nell'età più vulnerabile tutti i diritti: il diritto all'infanzia, al gioco, alla spensieratezza, all'istruzione la possibilità di scegliere, di amare, di decidere della propria vita e del proprio corpo; schiave di padri prima e di mariti dopo, e spesso anche schiave di suocere, cognate, donne che dovrebbero accompagnarle e aiutarle. La mozione di cui abbiamo discusso, e per la quale anch'io ringrazio molto la vice presidente Fedeli ricordando di averla sottoscritta, credo contenga le questioni davvero importanti e fondamentali. Approvando questa mozione noi chiediamo che siano promosse e rafforzate la tutela dei diritti e la parità di genere, i diritti umani delle donne e delle ragazze, il loro *empowerment* in tutti settori, il rafforzamento, la loro forza. Non si tratta unicamente, come è tuttavia fondamentale, che siano rispettati e sostenuti finanziariamente e politicamente gli impegni internazionali Il nostro Paese e il nostro Governo partecipano in maniera importante ai programmi internazionali di sostegno per il rispetto dei diritti delle donne e a quelli relativi a

Questa mozione chiede di più, un impegno politico e culturale per scardinare il principio secondo cui i diritti di una donna, di una bambina, di una minore, delle minoranze etniche valgono meno del diritto di altri. Questa mozione chiede che la politica scelga l'imperativo categorico dell'etica; chiede di continuare l'impegno internazionale per riuscire ad ottenere la fine di un fenomeno che imprime violenza sul corpo delle bambine e ne segna la vita per sempre, determinandone anche in molti, troppi casi, la morte. Chiede che non ci volgiamo dall'altra parte dinnanzi ai bambini nati da queste unioni violente, perché saranno uomini e donne di domani destinati ad una vita precaria ed infelice. Ancora di più chiede al nostro Paese di dotarsi di una normativa nuova che prenda atto che l'altrove oggi è qui. Una mozione che interpella le nostre coscienze e il nostro senso delle istituzioni e della politica come servizio alla società umana tutta.

colleghi, la seduta è ripresa. Il protrarsi della riunione del Consiglio di Presidenza, che è stato convocato convocato *ad horas* per decisioni da assumere, non ci consente di completare l'ordine del giorno. Quindi, in ragione di questa interruzione dei lavori della nostra seduta per la riunione che si è testé conclusa, i disegni di legge di ratifica di accordi internazionali saranno

*(Applausi).* Signor Presidente, faccio rilevare alla Presidenza che non è stata usata cortesia nei nostri confronti. avrei detto cose analoghe. Tuttavia, da parte mia personale e della Presidenza non c'era alcuna intenzione di ledere la dignità dei colleghi. Capita, a volte, anche nei lavori parlamentari, cui lei partecipa, che una seduta di Commissione che si protrae, un parere su emendamenti o una riunione del Consiglio di Presidenza determinino una variazione rispetto alle abitudini sue che so essere, negli ambiti in cui ha svolto i suoi

Signor Presidente, nell'area industriale di Pontedera, in provincia di Pisa, i lavoratori della società Iscot sono rimasti per quasi un mese in presidio fuori dai cancelli

che vengono rinnovati sotto la minaccia della perdita del posto di lavoro. Sono costretti, quindi, ad accettare tutte le condizioni dettate dall'azienda nella speranza di avere il periodico rinnovo contrattuale. La situazione a Pontedera è incandescente e rappresenta un modello di precarizzazione del lavoro e sfruttamento ormai diffuso in tutto il territorio nazionale. Molti sono gli interinali che subiscono vessazioni e troppi sono i casi di mancata denuncia e assenza di controllo preventivo. Dove è l'ispettorato del lavoro, che dovrebbe prevenire e disinnescare sul nascere queste situazioni? Dove sono i principali sindacati? I lavoratori lamentano l'assenza delle istituzioni che al loro posto lasciano spazio alle Forze dell'ordine che schedano i manifestanti. Tali lavoratori sarebbero stati costretti a lavorare per sette mesi con turni massacranti, sopportando provocazioni continue assimilabili al *mobbing*. Vessazioni e sfruttamento continui hanno portato i lavoratori della Iscot a intraprendere una battaglia per i loro diritti. La protesta che li ha condotti a presidiare i cancelli della Sole SpA ha richiamato l'attenzione dei *media* e dell'opinione pubblica. Ricordo che l'azienda Sole, Sole, che è stata interpellata e non risponde, è del vice presidente di Confindustria Maurizio Stirpe. L'azienda sembrava aver compreso le motivazioni della contestazione e il 22 settembre ha convocato i lavoratori per firmare sette contratti a tempo indeterminato, accogliendo le loro richieste. Tuttavia, l'azienda ha poi fatto marcia indietro, richiamando due degli operai, tra i più attivi nel difendere i propri diritti, informandoli che non potevano più prestare servizio sull'appalto perché la società Sole SpA li aveva identificati come soggetti in grado di turbare l'organizzazione del lavoro in azienda. È un caso gravissimo. Nella giornata dell'8 ottobre 2016 c'è stata una nuova lacerazione: un tentativo da parte dell'azienda di sostituire in blocco i lavoratori con nuove maestranze, che si sono presentate ai cancelli, fatto fermamente denunciato e respinto da parte dei lavoratori. Il lavoro non deve trasformarsi in una forma di schiavitù: lo denunciamo tutti i giorni, in Aula e nella Commissione lavoro. È grave che contratti sempre più flessibili e con scarse tutele vengano usati come forma ordinaria per l'assunzione di personale nelle aziende. Il lavoro interinale serve, evidentemente, per avere lavoratori usa e getta

Proprio per questo ho depositato un'interrogazione al ministro Poletti, affinché il Ministero del lavoro intervenga immediatamente su questa situazione gravissima. Da parte mia e del Gruppo Movimento 5 Stelle diciamo ai ragazzi della Iscot che siamo a loro fianco: resistete, resistete, resistete!

Grazie,